L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,

senatore Tonini con una sottolineatura, che avevamo già fatto nella precedente lettura, sui tempi delle ratifiche: un tema non nuovo, ma ormai strutturale del nostro sistema.

un Accordo fatto il 3 giugno del 2002 che viene ratificato quasi dieci anni dopo non onora il nostro Paese e, soprattutto, è un chiaro segnale di inefficienza della nostra struttura amministrativa. Non è ovviamente una responsabilità che attribuiamo a questo Governo in particolare, perché è una lunga e non gloriosa tradizione del nostro Paese quella di impiegare così tanto tempo per le ratifiche. Sollecitiamo in ogni caso a mettere in atto qualche provvedimento, istituendo magari una commissione che studi modalità più rapide per ottenere il concerto dei Ministeri: condizione essenziale, questa - una volta accelerato, come siamo riusciti a fare, l'*iter* parlamentare

In Commissione il provvedimento è stato approvato all'unanimità. Esso, ripeto, ha una sua importanza perché ribadisce anche la sede del Segretariato esecutivo a Trieste, attraverso anche uno snellimento dell'organigramma. Quindi, il provvedimento è positivo ed invito ad approvarlo.

del Gruppo del PD. Mi preme soltanto significare alla vostra attenzione l'importanza che assume la collocazione del Segretariato esecutivo dell'InCE nella città di Trieste. È una scelta frutto della stessa importante collaborazione garantita dalla regione Friuli-Venezia Giulia, di cui Trieste è capoluogo, ma ritengo sia anche un giusto e doveroso riconoscimento ad un'area del Paese che da sempre, e la sua storia lo insegna,

Signora Presidente, anche questo è un provvedimento di importanza notevole. Esso va a rafforzare la cooperazione culturale tra Italia e Siria, aumentando le attività già previste in un precedente Accordo bilaterale risalente al dicembre del 1971. del 1971. L'Italia e la Siria si trovano ad un ottimo livello di rapporti diplomatici, anche grazie ad aperture che il Governo di Damasco ha attuato ultimamente nel dialogo verso l'Occidente. da questo punto di vista, questo provvedimento assume oggi una sua rilevanza, oltre che per il considerare il terreno delle culture come assolutamente privilegiato per instaurare maggiori rapporti e portare

completamente diverso ma, purtroppo, non è necessariamente diverso il regime che governa la Siria, Paese che, ricordiamolo, è una Repubblica che si definisce araba, e già questa sua questa sua aggettivazione, in qualche modo, mette in evidenza alcuni problemi che poi si sono venuti ad articolare con il passare del tempo. Tali problemi si stratificano con il passare degli anni, ma partono già dagli anni Sessanta, quando è stata imposta una sorta di legge marziale o, comunque, una serie di leggi emergenziali che pongono sotto tutela qualsiasi tipo di libertà. Essendo il nostro un trattato

(va detto che la Siria, malgrado la popolazione non goda necessariamente né di libertà, né di pieni diritti economici e sociali, sicuramente non è tra i Paesi più poveri al mondo) poveri al mondo) per preservare un patrimonio culturale che appartiene a tutta l'umanità poiché conserva parti importanti di culture non soltanto mediorientali, ma anche fondative della nostra comunità

all'articolo 16 prevede le modalità per denunciare lo stesso (cosa che invece, per esempio, non è avvenuta con l'Accordo bilaterale Italia-Libia) - parla di cooperazione culturale e, oltre al settore archeologico e artistico, auspica il rafforzamento della collaborazione tra le università e tra gli archivi nazionali dei due Paesi, e addirittura arriva ad auspicare un rafforzamento della collaborazione in materia di audiovisivi, quindi documentari e

anche quelli che hanno avuto da ridire non soltanto sugli atteggiamenti politici siriani a livello nazionale, ma anche sul coinvolgimento della Siria

l'occupazione, anche militare, della Siria nei confronti del Libano, cessata qualche anno fa, e non perché sia stato liberamente scelto da Damasco di ritirarsi, ma perché, a seguito dell'omicidio del già premier libanese Rafik Hariri, e degli interventi e delle insistenze della comunità internazionale (Francia, Regno Unito e Stati Uniti, *in primis*), e poi dell'apertura delle indagini per la ricerca dei responsabili dell'omicidio stesso, la Siria ha deciso di diminuire (perché credo non si possa oggi certificare la totale assenza di militari siriani dal Libano) la propria presenza nel Paese vicino. L'altra grande alleanza storica, che credo preoccupi tutti coloro i quali hanno a cuore, oltre la stabilità anche la pace e la libertà del Medioriente, è quella con il regime di Teheran, che da sempre utilizza la Siria per allungare i propri tentacoli verso il Mediterraneo, e che sta anche "invadendo" dal punto di vista economico, oltre quindi che culturale, un Paese a maggioranza sunnita, ma governato da una minoranza sciita. Amnesty International ci ricorda, per esempio, che il modo con cui viene amministrata la giustizia è totalmente al di fuori dei canoni internazionali, perché viene praticata la tortura per una serie di crimini tra i quali, ripeto, sono ricompresi Ci sono enormi problemi per quanto riguarda le minoranze (per esempio, quella curda), ma altrettanti problemi riguardano la minoranza palestinese rifugiata in Siria; le donne non hanno gli stessi diritti che vengono riconosciuti agli uomini. I profughi che fuggono dall'Iraq o dall'Iran, anche se si tratta di arabi (per esempio, gli ahwazi che fuggono dalle persecuzioni iraniane e che il Senato della Repubblica italiana ha potuto audire nel maggio scorso presso la Commissione straordinaria per a un trattamento che va ben oltre quello che anche noi, alle volte, riserviamo ai cosiddetti immigrati clandestini, e sono a forte rischio di deportazione o respingimento.

In due occasioni, nel dicembre 2008 e nel dicembre 2010, la Siria, che appunto continua ad applicare la pena di morte, ha votato contro la proposta di risoluzione italiana a favore della

anche con regimi che si discostano dalla pratica della democrazia e sui quali la comunità internazionale ha assunto deliberazioni formali di netta denuncia della sistematica violazione dei diritti fondamentali»

i diritti umani), il Senato ritiene che vadano subordinate «tali relazioni agli obblighi internazionali derivanti all'Italia dall'aver ratificato tutti gli strumenti internazionali sui diritti umani» (un principio, questo, che credo debba rimanere guida della nostra politica internazionale), si chiede al Governo di assumere un impegno «a sostenere ogni accenno di annunciato impegno in riforme politiche ed economiche, e a favorire l'affermarsi di tale posizione anche a livello europeo, al fine di migliorare la propria credibilità verso l'integrazione regionale e internazionale, con particolare attenzione anche alle voci di chi, istituzionalmente, non partecipa al processo decisionale preclusogli da un regime non democratico; a promuovere e favorire ogni azione, a livello europeo ed internazionale, tesa ad assicurare che la Siria disponga una moratoria delle esecuzioni capitali e avvii una profonda revisione del codice penale, rendendo più accessibile, oltre che da entità ufficiali delle Nazioni Unite

sia autoctone sia che risultino presenti, per ragioni diverse, in Siria, e conseguentemente ad attivarsi al fine di favorire il rispetto delle prerogative tradizionali e culturali di tali minoranze oltre ai diritti fondamentali universalmente riconosciuti, nonché i casi di denegata giustizia raccolti da numerose organizzazioni internazionali sui diritti umani.

la ratifica dell'Accordo in esame credo che incontri il consenso unanime del Senato, così come è avvenuto alla Camera.

Il ministro Frattini è stato di recente proprio in Siria, e noi stiamo monitorando con particolare attenzione l'evolversi della situazione in quel Paese, alla luce di quanto avviene in tutta la regione. Per questi motivi, sulla base di queste brevissime considerazioni, venendo all'ordine del giorno, il Governo, tralasciando la valutazione sulle motivazioni, che attengono a

coincidendo sostanzialmente la posizione espressa nell'ordine del giorno con quella che il Governo sta seguendo sul campo.

con il parere espresso dal Governo, e ricorda che questo provvedimento è stato approvato all'unanimità dei presenti in Commissione proprio il giorno in cui il Ministro degli affari esteri ha visitato la Siria

la cultura, essendo l'Italia e la Siria (l'Italia nel mondo e la Siria tra i Paesi mediorientali) gli Stati che hanno il maggior numero di

favorevole del Gruppo del Partito Democratico, motivato dalla valenza strategica della Siria, che è un Paese assolutamente cruciale del Medio Oriente.

In particolare, il tema della cooperazione culturale è forse il canale migliore e più giusto per intraprendere queste relazioni. Proprio per questo, però, l'esperienza, tanto più di queste settimane, ci insegna che non è pensabile un'amicizia con Paesi importanti come quelli arabi, con i quali l'Italia ha una tradizione lunga di relazioni attente e positive, che escluda dalla sua attenzione il tema dei diritti umani. il necessario rispetto per il percorso di ogni Paese e per la sua sovranità, è importante che l'Italia, nello stabilire relazioni positive con questi Paesi, non dimentichi mai la dimensione essenziale dei diritti umani. Anche per questo motivo, abbiamo sostenuto l'ordine del giorno proposto dal collega Perduca, che ringraziamo per il suo importante contributo su questo passaggio. Insieme a tale ordine del giorno, è con questo spirito che votiamo a favore della ratifica.

pubblicato in data 20 ottobre 2010. Si tratta, signora Presidente, di un lavoro piuttosto complesso, un'interrogazione che abbiamo rivolto al Ministro del lavoro ricostruendo

cui purtroppo è corrisposto peraltro, parallelamente, anche l'incremento delle liste di mobilità e di disoccupazione. Chiediamo al Ministro di sapere se le aziende beneficiarie di questo ingente volume di erogazioni per la cassa integrazione straordinaria abbiano ora normalizzato il processo produttivo, e quali iniziative il Governo intende promuovere per arginare la crisi economica che vive il mondo delle imprese in Piemonte che, data la sua ampiezza, l'entità delle risorse, il numero degli addetti e il peso nel PIL nazionale, e considerata la vocazione manifatturiera della Regione, se non governata avrà effetti di lungo periodo sulla vita economica del Paese. Si tratta, vale a dire, di un'analitica ricostruzione di tutti i provvedimenti di cassa integrazione straordinaria, e chiediamo, appunto,

che riguardano una delle questioni più importanti in merito alle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, dicembre 2005, n. 262, che all'articolo 19 stabiliva l'adozione di un regolamento per definire gli assetti proprietari di Bankitalia e le sue modalità di trasferimento entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. Entro il 28 dicembre 2008 il Governo doveva quindi stabilire un regolamento per sottrarre l'istituto di vigilanza Bankitalia di Mario Draghi alle grinfie delle banche. Ciò non è avvenuto, e lei comprenderà, signora Presidente, e lo comprenderanno anche i colleghi, che tale questione è importante. Faccio questo intervento all'indomani della richiesta,

chiedono un "pizzo" di tre euro: hanno inviato una lettera dove richiedono tre euro per prelevare il contante allo sportello.

milioni di risparmiatori truffati dalle banche e dagli omessi controlli di Bankitalia.

L'anno scorso abbiamo discusso il nostro bilancio a settembre: un bilancio che, ricordo, è preventivo e non consuntivo. Credo che, prima di passare alla non violenza per avere quello che ci deve essere dato per tempo, occorra avere dalla Presidenza informazioni certe circa la distribuzione del documento, sul quale dovrà essere dato poi ai senatori il tempo necessario per avanzare i propri rilievi. **Per

portatore della sua fede cristiana. È una cosa che non ci fa certamente onore, mentre i giornali ancora una volta parlano dell'allontanamento del crocefisso